comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente convocata per domani, giovedì 13 novembre 2008, alle ore 9, per procedere alla propria costituzione. Onorevoli colleghi, è per il Senato un momento solenne ricordare, in occasione dei cento anni dalla nascita, Giovanni Leone, già nostro collega, figura di primo piano nella vita istituzionale del Paese, uomo dalle grandi doti umane e civili. Giovanni Leone nacque a Napoli il 3 novembre del 1908. Ricordare le tappe della sua vita significa ripercorrere quasi un secolo di vicende della storia e della politica italiane, a cominciare da quando a Napoli, avvocato e studioso di diritto e procedura penale, cominciò a militare con passione politica e civile nell'Azione cattolica. Si impegnò allora, in clandestinità, per un'Italia democratica che portasse il Paese fuori dal regime fascista, riprendendo il filo della partecipazione popolare attraverso i grandi partiti e contribuendo in quest'ottica alla nascita della Democrazia Cristiana. Eletto il 2 giugno 1946 deputato all'Assemblea costituente,

Il prezioso contributo del giurista Giovanni Leone nelle aule della Costituente gli valse il prestigio e un'autorevolezza tale da portarlo a ricoprire la carica di Vice presidente della Camera dei deputati nel 1950 e nel 1953 e quindi, nel maggio 1955, ad essere eletto Presidente di quel ramo del Parlamento. Carica, questa, confermata poi nella III e IV legislatura. Anche in questo ruolo seppe distinguersi per equilibrio, offrendo le sue doti di guida e mediazione nella direzione delle discussioni parlamentari in un periodo di grandi contrapposizioni politiche. Con questo stesso spirito affrontò i successivi incarichi di Governo negli anni Sessanta, impegnandosi a favorire il dialogo tra democristiani e socialisti, in un'ottica che aveva come fine primario il mantenimento di un ordinato clima politico che potesse poi eventualmente garantire equilibri diversi fra i partiti. Il 24 agosto del 1967 è nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat per altissimi meriti in campo scientifico e sociale, un riconoscimento a Leone maestro del diritto, che precede di pochi anni il raggiungimento da parte sua del gradino più alto delle nostre istituzioni, con l'elezione a Presidente della Repubblica il 24 dicembre 1971. Le sue parole nel discorso di insediamento ribadirono il compito che nella sua visione costituzionale la massima carica doveva svolgere: vigilare sull'osservanza della Costituzione e promuovere il buon funzionamento dei congegni costituzionali, tenendosi al di fuori dei difficili equilibri politici del momento. Il periodo della presidenza Leone fu infatti tra i più complessi della storia politica italiana, caratterizzato da profondi cambiamenti nella società e da avvenimenti drammatici che colpirono profondamente l'intero Paese. Tale periodo fu accompagnato da una forte instabilità del quadro politico ed elettorale e negli stessi anni si assistette ad un inasprimento dei conflitti sociali e all'offensiva del terrorismo e dello stragismo, in una spirale di violenza sempre più cieca, culminata con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro nel 1978. Furono, questi, giorni di dolore e di incertezza per il Paese e il presidente Leone si adoperò per contribuire ad una soluzione che non fosse quella, poi drammaticamente verificatasi, dell'uccisione dello statista. La fine tragica di quella vicenda determinò l'impossibilità di ricomporre il quadro politico e segnò l'inizio della fase finale della cosiddetta prima Repubblica. In questo contesto, lo stesso Leone pagò un prezzo altissimo: dimessosi dalla carica, fortemente amareggiato, tornò a dedicarsi agli studi ed alla ricostruzione puntuale, in tutte le sedi, delle vicende drammatiche di quegli anni. Del presidente Leone ricordiamo oggi lo spirito di dedizione allo Stato repubblicano, il senso di equilibrio, il rigore sempre accompagnato da grande umanità, la lunga attività politica in difesa della democrazia e dei diritti individuali e collettivi, la passione - che lo accompagnò fino alla fine - per il diritto. Prima di concludere, voglio ricordare l'impegno del Senato per conservare la documentazione del Fondo Leone; l'Archivio storico ha intrapreso l'opera di ordinamento ed inventariazione analitica del Fondo, che copre l'arco cronologico compreso tra gli anni Venti e il 2001. Il Fondo comprende lettere, discorsi, articoli ed interviste, documenti e questioni relativi all'attività istituzionale, nonché a quella di docente universitario e avvocato, insieme alle memorie dettate dal presidente Leone ai suoi collaboratori nel corso della sua vita e a numerosi album fotografici, cassette audio e video. Di tale rilevante contributo all'Archivio storico del Senato ringraziamo sentitamente la famiglia. Ed alla famiglia, sempre punto centrale della sua esistenza e a lui sempre vicina, certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, rinnovo oggi il nostro saluto affettuoso e commosso.

un uomo che ha dedicato la propria vita alla concretezza degli ideali, una figura emblematica della storia della nostra Repubblica; costituente, deputato e senatore ma soprattutto, almeno per noi, giurista di chiara fama e, infine, grande Presidente della Repubblica. Grande giurista il presidente Leone; chi, come noi, ha studiato i suoi libri, a cominciare dal manuale di procedura penale, può apprezzare forse ancora di più la veste di questo insigne padre della Patria e può apprezzare il contributo da lui dato alla storia repubblicana da giurista e da cultore della Costituzione prestato alla politica, quale secondo noi egli è stato, il contributo che lui ha dato con grande impegno alla crescita delle istituzioni italiane. Non credo sia necessario ricordare i passaggi importanti, perché lo ha già fatto lei, della vita di di Giovanni Leone. Certamente a noi preme sottolineare alcuni aspetti che sono importanti: primo tra tutti la circostanza che per Leone la politica non era un mestiere. Egli non era un politico di ruolo ma molto di più, perché aveva un impegno morale ed etico superiore a ciò che ciascuno potesse immaginare. E dedicò alla politica come missione tutta la sua vita portando nelle istituzioni quella sua profonda e grande cultura giuridica e giuridica e costituzionale che troviamo, ad esempio, anche e soprattutto nella parte relativa alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura, che fu la parte di cui egli si occupò quando fu eletto alla Costituente. L'altra considerazione che a noi piace fare sulla vita e sull'attività di Giovanni Leone è quella che ha segnato il suo settennato di Presidente della Repubblica. Un settennato che lui ha interpretato con il ruolo tradizionale e discreto del Capo dello Stato; un settennato nel quale ha dimostrato di avere una grande capacità anche di mediazione e di risoluzione di controversie che riguardavano la contesa politica di quegli anni, a cominciare dalla elezione dei primi giudici costituzionali. Un settennato contrassegnato anche dalla triste vicenda del caso Moro e del ruolo che anche sotto il profilo umanitario oltre che istituzionale il presidente Leone ha svolto in quel periodo, e che è tutto da approfondire e da studiare anche oggi, a distanza di 30 anni dall'eccidio di via Fani. Credo sia giusto in questo momento, anche al di là della retorica di questi momenti particolari e cerimoniali, fare una considerazione che può apparire un po' fuori dalle righe. Le dimissioni del presidente Leone suscitarono allora grande scalpore e furono il frutto di una campagna mediatica di pessimo gusto e di profondo squallore, che lui visse con grande sofferenza, ma che lo portò, con grande dignità, a dimettersi, uscendo dalla scena politica senza grossi clamori, in punta di piedi, portando con sé una profonda malinconia, convinto di essere vittima di un'ingiustizia, così come la storia ha accertato, fidando con fatalismo tutto meridionale nel tempo che, a volte, sa essere galantuomo. Riteniamo che il tempo sia stato galantuomo con il presidente Leone e che alcuni personaggi protagonisti allora della campagna di delegittimazione del presidente Leone nel tempo gli abbiano chiesto scusa. Mancano all'appello ancora alcuni, che dovrebbero chiedere scusa a questo grande democristiano che ha fatto la storia e le istituzioni di questo Paese. Riteniamo sia giusto oggi ricordarlo come merita e la ringraziamo per ciò che lei, come Presidente del Senato, ha fatto e sta facendo perché la storia di Giovanni Leone sia ascritta alle pagine migliori della storia repubblicana italiana.

Mi emoziona farlo perché anch'io, come intere generazioni - e molti siedono in quest'Aula - mi sono formato sui libri di Giovanni Leone, sul suo manuale di diritto processuale, che dal 1960 divenne il testo adottato da quasi tutte le università italiane; considerato maestro da tutti, lui, che era stato l'allievo prediletto di Enrico De Nicola. Mi piace ricordare che la sua tesi di laurea ebbe come argomento la violazione agli obblighi di assistenza familiare; era una tesi sperimentale, perché quella norma ancora nel nostro codice Rocco non c'era; lui si ispirò al diritto francese

anni scrisse un libro fondamentale sul reato continuato, sul reato abituale e sul reato permanente, libro che rimane tale; a

Fu all'inizio un conoscitore e uno studioso del diritto penale sostanziale. Poi, in un periodo in cui la disciplina del diritto penale sostanziale era unificata a quella del diritto penale processuale, perché la cattedra era unica e quindi unico l'insegnamento, partecipò al concorso con un testo di diritto processuale. Da quel momento iniziò la sua enorme produzione di diritto processuale, attraverso i manuali, per arrivare poi a questa opera monumentale che è stata ed è il trattato di diritto processuale penale. Non amava il nuovo codice, quello che è entrato in vigore nel nostro Paese nel 1989; esso non era amato e non era apprezzato da Giovanni Leone, che era riuscito a capirne alcuni profondi limiti, quelli dei quali noi ci siamo accorti nel corso degli anni. Eppure, la sua critica non riuscì, se non limitatamente, a produrre risultati perché ormai cominciava ad essere stanco nella sua produzione.

la Corte di cassazione che, in tema di diritti della difesa, riteneva che quei diritti si applicassero all'istruttoria formale e non all'istruttoria sommaria. Fu una battaglia fondamentale, che si concluse poi con la vittoria di quei principi, tant'è che la Corte costituzionale dovette intervenire. Da lì cominciò il processo moderno con i diritti della difesa; arriveremo al giusto processo, ma fu da quella battaglia condotta da Giovanni Leone che cominciarono a concretizzarsi i diritti della difesa nel processo penale. Io ritengo che debba anche ricordarsi un suo cruccio, la sua voglia di poter cambiare anche il codice penale, che egli riteneva superato. In quest'Aula, egli fu relatore per la riforma del codice penale: il progetto Gonella del 1968 proprio in quest'Aula vide protagonista Giovanni Leone. Poi quel progetto si arenò, come tutti gli altri progetti che seguirono, ma egli aveva comunque visto la necessità di intervenire sul codice penale del 1930 e rimase un suo cruccio non aver potuto vedere la realizzazione di questo suo sogno.

rimane consacrata negli atti da lui compiuti che lei, signor Presidente, ha qui ricordato

anche noi del Gruppo della Lega Nord ci associamo e condividiamo le parole espresse dal presidente Schifani ringraziamo la Presidenza di questo Senato per aver voluto ricordare in questo momento la figura di Giovanni Leone, è stata una delle più discusse della storia politica italiana. La sua Presidenza della Repubblica, scaturita dopo oltre 20 votazioni con una manciata di voti, è stata purtroppo attraversata da scandali e da accuse che lo costrinsero alle dimissioni. Ad ipotecare, se non ad inquinare, la sua elezione furono i voti decisivi dell'allora Movimento Sociale Italiano. Poi la vicenda della Lockheed, che lo mise in ginocchio e per la quale fu riabilitato solo vent'anni dopo: immaginate le sofferenze dell'uomo, in una situazione del genere. Fu anche Presidente del Consiglio di quel Governo che fu definito balneare per la sua durata stagionale, e fu apprezzato Presidente della Camera, com'è già stato ben ricordato. Oggi, a cento anni dalla sua nascita, occorre menzionarne la statura di giurista ed avvocato, in cui la cultura ben si sposava con l'acuta intelligenza e quella fervida vivacità napoletana che lo vide protagonista negli storici processi in tutta Italia. Il senatore Li Gotti ha ricordato che sui suoi testi di procedura penale hanno studiato e si sono formate generazioni di studenti, conquistati dalla sua chiarezza scientifica ed espositiva. Fu tra i padri della Repubblica e giocò un ruolo importante nella scrittura della Costituzione;

e che ne sminuirono il personaggio e la figura, di assoluta caratura professionale e politica. Ma la sua *verve*, il suo ottimismo e le sue battute furono smorzati dalle vicende che travolsero lui e la sua famiglia, anche soprattutto per la campagna che il settimanale «L'espresso» condusse contro di lui, senza esclusione di colpi. Ma oggi lo ricordiamo con la nobiltà del tempo, che si è rivelato galantuomo con lui gli ha dato da morto quello che gli aveva tolto in vita. Riposi in pace, professor Giovanni Leone! Signor Presidente, desidero associarmi, a nome mio personale e del Gruppo che rappresento, al ricordo espresso in quest'Aula del presidente Giovanni Leone. Nel farlo, vorrei cominciare dalla fine della vita pubblica dell'ex Presidente, da quella sera drammatica del 15 giugno 1978 quando, alle ore 20,10, si affacciò sugli schermi televisivi per il suo ultimo messaggio agli italiani, dicendo: «Non v'è in me il rimpianto di lasciare questa carica, ma rimpianto grave sarebbe quello di lasciare in voi un'ombra di sospetto sulla suprema istituzione della Repubblica. Credo che oggi oggi abbia io il dovere di dirvi - e voi, come cittadini italiani, abbiate il diritto di essere da me rassicurati - che per sei anni e mezzo avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto, che ritiene di aver servito il Paese con correttezza costituzionale e dignità morale»*.* Non solo per noi che oggi lo onoriamo, ma da tempo queste tre doti di Giovanni Leone (l'onestà, la correttezza costituzionale e la dignità) gli sono riconosciute unanimemente; anche se non manca, tra coloro che ne favorirono o ne vollero allora la caduta, chi ancora si attarda in giustificazioni o imbarazzati silenzi. Ma quella sera drammatica il presidente Leone disse, proprio in chiusura, anche un'altra cosa che dimostra un'ulteriore sua dote, quella dell'intuizione, che precede l'intelligenza e la comprensione dei fenomeni. Parlando non più a difesa sua, ma di tutti i cittadini, delle nostre istituzioni e della corretta vita democratica, disse: «Sono certo che la verità finirà per illuminare presente e passato e sconfessare un metodo che, se mettesse radici, diventerebbe uno strumento fin troppo comodo per determinare la sorte degli uomini e le vicende della politica». Giovanni Leone è stato una figura emblematica della storia della Repubblica: costituente, deputato, senatore, giurista di chiarissima fama e, infine, Presidente della Repubblica. La sua ascesa e la sua eclissi fanno parte di un periodo storico in cui la Democrazia Cristiana era padrona assoluta della scena politica. Come giurista lavorò a fianco di De Nicola e di Francesco De Martino; come docente universitario ebbe tra i suoi assistenti Aldo Moro. Con i suoi studi monografici e con i suoi trattati fu maestro in Italia e all'estero di generazioni di studenti e di studiosi. Questa passione, questa competenza giuridica egli portò in politica quando alla fine della guerra, sulle orme del padre che fu tra i fondatori del Partito Popolare, entrò nella Democrazia Cristiana. La sua straordinaria competenza giuridica fu unanimemente apprezzata sin dalla Costituente dove, divenuto membro della Commissione dei 75, dette il meglio di sé sulle questioni riguardanti l'ordinamento della magistratura. le sue intuizioni si rivelarono giuste e lungimiranti: quando si impegnò a difesa dell'ordine giudiziario per la istituzione del Consiglio superiore della magistratura, come quando si batté per la separazione del ruolo dei magistrati giudicanti da quelli requirenti che egli vedeva, come accade nella maggior parte degli ordinamenti continentali, espressione del potere punitivo dello Stato.

Da un punto di vista politico e giuridico, come hanno ricordato molti insigni giuristi e uomini politici, il settennato del presidente Leone fu perfettamente corretto. Si cercò di imputargli il coinvolgimento in alcuni scandali pubblici sulla base di argomenti del tutto infondati che mai trovarono prova di ciò, anche se a distanza di anni, tutti o quasi gli accusatori di allora - a cominciare da Marco Pannella - chiesero scusa all'ex Presidente. Tutto ciò - disse il presidente Leone a commento di queste tardive scuse dimostra che non sempre è necessario dover aspettare la conclusione di una vita per restituire dignità e onore a chi ha sempre operato con correttezza. Parole dalle quali tutti noi dovremmo trarre insegnamento, tanto più in un momento come quello attuale in cui sentiamo il bisogno di una politica che, pur affermando i suoi ruoli di appartenenza, deve essere capace di interpretare il bene comune e un senso di responsabilità alto verso le istituzioni e verso il Paese. Commemorare significa ricordare insieme, ma le commemorazioni rappresentano anche un rischio perché racchiudono il significato della vita di una persona in una gabbia di parole che non rappresentano interamente quella persona, ma solo ciò che noi, spesso arbitrariamente, vogliamo conservare di lui. Ecco, se dovessimo sintetizzare, l'interesse generale e il bene comune sono stati i fondamenti dell'azione politica di un grande uomo italiano che oggi anche qui in Senato vogliamo ricordare non solo con affetto, ma anche con la gratitudine che si deve a chi ha contribuito a rendere questo Paese democratico.

Giovanni Leone fu una figura politica e istituzionale cruciale di quella che, con un certo arbitrio, ci ostiniamo a chiamare prima Repubblica, come se nel frattempo avessimo davvero costruito la seconda. Figura politica e istituzionale, ma molto più istituzionale che politica, ebbe un ruolo centrale nella vita dello Stato e un ruolo molto più periferico negli equilibri del suo partito. Scalò grado a grado le vette della Repubblica: fu Presidente della Camera, Presidente del Consiglio, Capo dello Stato. Non fu *leader* politico, non fu figura di parte, non ebbe mai dalla sua il sostegno di gruppi organizzati, di tessere di partito, di correnti, tanto meno di clientele. Questa fu la sua debolezza ma credo anche, in qualche modo, il suo orgoglio; in ogni caso, fu la sua cifra. Era un uomo all'antica, custode di un'Italia tradizionale, che con la democrazia e con il miracolo economico stava cambiando pelle. Un grande avvocato, un maestro di diritto, tenacemente legato ai suoi studi e alla sua professione. Un uomo, se così si può dire, più figlio dell'Ottocento che padre del Novecento, più legato al misurato e prudente notabilato cattolico e liberale dell'Italia del Sud, che alle smisurate, eccessive ideologie del secolo breve finito nel 1989. Oggi ricordiamo il primo centenario della nascita e l'occasione celebrativa induce a ricordi dolci e non troppo controversi, ma faremmo un esercizio di ipocrisia - e non lo hanno fatto i colleghi intervenuti prima di me se nascondessimo a noi stessi la ferita di quella controversia profonda che lo portò alle dimissioni prima del tempo. Negli ultimi anni del suo settennato presidenziale, Giovanni Leone fu oggetto di un'aggressione politica e mediatica che lasciò il segno, un'aggressione da cui Leone si può dire che quasi non si sia difeso, opponendovi più la sua incredulità, che non le sue prerogative politiche e presidenziali. Le sue dimissioni furono il primo evento che si produsse nella nostra vita pubblica all'indomani dell'assassinio di Moro, e tutto avvenne in modo così lacerante, credo anche per il venir meno di quell'accorta regia negli equilibri del Paese di cui Moro, più di tutti, si era dimostrato capace in quegli anni. All'indomani della sua uscita dal Quirinale, Leone votò per Pertini, un uomo politico e un Presidente tanto diverso da lui; si iscrisse al Gruppo Misto e qualche anno dopo rientrò in punta di piedi nel Gruppo del suo partito. Se ebbe delle amarezze, riuscì a non trasformarle mai né in rancori, né in veleni, e anche in questo si può ravvisare una cultura delle istituzioni che, da allora ad oggi, si è un pochino dispersa. In quegli anni la sua famiglia fu la sua tana e la ragione del suo compiacimento. Non si tratta oggi, a distanza di tanto tempo, di ripercorrere dopo passo quella vicenda; semmai si può segnalare che molti di coloro che furono in prima fila nell'animare quella campagna contro il Quirinale, anni dopo sono stati altrettanto in prima fila nel capovolgerne valori e significati. Il destino di Giovanni Leone è stato, in fondo, quello di tanti democratici cristiani, avversati con durezza negli anni della gloria e rivalutati, perfino rimpianti, dai loro avversari di una volta, quando quella gloria poi è finita. Ogni figura che ha lasciato un segno nella vita pubblica del Paese deve rassegnarsi ad accettare la controversia ed anche certe asprezze che la accompagnano; ma un grande Paese, a sua volta, deve essere in grado di ricucire le sue ferite, di chiudere le sue controversie e restituire alle sue figure più significative l'onore politico che non avevano mai perduto. Credo che faccia bene alla Repubblica ricordare uno dei suoi Presidenti come un uomo di valore che ha servito il proprio Paese in anni non facili come meglio poteva, con quella lealtà repubblicana che lega i padri e i figli, e che riguarda il nostro tempo non meno di quello che è toccato in sorte a Giovanni Leone.

Signor Presidente, nel 1978, all'indomani del dramma di Moro, a qualcuno parve che Leone potesse prestarsi a diventare un Capo dello Stato ricattabile. Di fronte alla sola ipotesi, Giovanni Leone preferì dimettersi, pur di non destare un'impressione del genere. Il diritto al «non ci sto» volle precluderselo con estrema fermezza

la campagna diffamatoria sembrava aver intaccato la fiducia delle forze politiche e che la sua scelta non poteva che essere quella,

ha iniziato, al principio degli anni Sessanta, una critica alla cosiddetta partitocrazia meno retorica, ma non meno efficace, di quella dei Maranini e dei Sartori, per restare nell'ambito accademico, o di quella degli Jemolo o dei Pacciardi, per far riferimento al dibattito più generale delle idee. In Leone quella scelta fu dettata da fedeltà alla Costituzione, allo Stato, al diritto: era la convinzione dolorosa, sofferta, ma nitida, di dover opporre alla bassezza di uomini e cose di quel periodo null'altro che la fedeltà alla propria vita, alla propria storia, alla propria Patria. Per lui, allora, lo ricordò Marcello Pera in chiesa all'indomani della sua scomparsa nel 2001, si aprì una silenziosa eppure orgogliosa stagione, la stagione nella quale ci si trova in quella zona grigia ai confini tra i tempi per loro natura ingenerosi della politica e quelli altrettanto ingiusti talvolta delle procedure del diritto. A Leone il proprio Paese chiese di voler più bene allo Stato che a se stesso. A suo modo era una richiesta con aspetti odiosi, ma ad essa Leone scelse di rispondere con quell'altissima idea dello Stato nazionale e della Patria costituzionale nella quale credeva e aveva saputo insegnare a credere alla generazione dei frequentatori dei suoi libri. Il Capo dello Stato, secondo Leone, è prigioniero della sua posizione e come tale è più debole ed indifeso di qualunque altro uomo politico. Ricorderà Giovanni Leone a Pietro Chiara, un uomo che gli fu assai più vicino, con sensibilità, di tanti altri, non poteva presentarsi e difendersi in Parlamento, perché era fuori dai suoi poteri e dalle sue prerogative costituzionali, né poteva emettere volta per volta una dichiarazione televisiva (le cosiddette esternazioni), perché il Presidente si doveva avvalere di tale mezzo solo per messaggi al Paese. Queste sono Altro che basso profilo! Quello della sua Presidenza fu il profilo del diritto, del ruolo di garanzia, mai di governo effettivo, che il Presidente della Repubblica deve sempre e comunque rappresentare e di cui gli avrebbero dato atto anche avversari politici: ricordo quando i radicali consegnarono a Leone la ricerca sugli atti della sua Presidenza coordinata da un grande giurista e un grande amico di Giovanni e Vittoria Leone, il compianto Vincenzo Caianiello. La dignità del vertice dello Stato come garanzia di potere neutro era in Leone dottrina che risaliva al Risorgimento, alla monarchia costituzionale. Come giurista l'aveva appresa da Vittorio Emanuele Orlando, del quale Leone aveva scolpito nella sua memoria giovanile il discorso fatto a Napoli al principio degli anni Venti (Leone era con suo padre, il giovane popolare Mauro Leone) e che poi fu pubblicato su «Il Mattino» del 1923. Il succo

anch'essa, non meno della monarchia, necessità di risorse, di potere neutro, in alcuni momenti. Ecco perché Leone precluse a se stesso - credo non ci abbia mai pensato - l'esercizio del personale diritto al «non ci sto». Per quelli che come me hanno avuto 20 anni nel 1968, ma il 1968 non lo hanno fatto, due sono stati i maestri incontrati a cavallo fra le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche sui cui scritti e discorsi ci siamo formati: uno era Norberto Bobbio e l'altro Giovanni Leone, due grandi amici. Si erano conosciuti nel 1935 quando Leone, professore antifascista, aveva dato il benvenuto al giovane professore di filosofia del diritto, risultato in un concorso, sotto il profilo antifascista, assai più discusso; fra Leone e Bobbio c'era stata una staffetta qui in Senato in Commissione giustizia. Ebbene, rispetto alla memoria di queste due importantissime figure più passano gli anni e più mi accade che il primo, Bobbio, mi sembri, non voglio dire sempre più piccolo, ma sempre più tecnico per quella sua stessa straordinaria capacità di giocare con le definizioni e le dottrine; il secondo, Leone, che mi sembrava troppo tecnicamente giurista negli anni Sessanta, oggi mi appare sempre più grande, proprio per non essersi mai fatto strumentalizzare o asservire alle sue definizioni e alle sue stesse dottrine. Mi è capitata poi la strana avventura in Senato di trovarmi "collega" di entrambi e di avere oggi l'onore di ricordare Giovanni Leone a 100 anni dalla sua nascita. Ricordare Giovanni Leone significa ricordare l'ultimo grande di una certa idea della storia d'Italia, un'idea di cattolicesimo liberale. Ne parlavo prima con un suo grande amico, il senatore Pisanu, che si trova a cavallo tra la generazione di Giovanni Leone e quella di mio padre. Leone da questo punto di vista è una figura estremamente Per Leone l'espressione cattolicesimo liberale è un'espressione vera e seria, non uno schema giornalistico. la persona umana, la filosofia del diritto di Giuseppe Capograssi, ma anche tutta la tradizione della destra storica, di Minghetti, di Arcoleo, nonché una conciliazione tra cattolicesimo e liberalismo, anche dello stesso Alessandro Manzoni. Rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto non mi sento di attribuirlo tutto e soltanto alla tradizione repubblicana. Vi sono molti istituti monarchici che Leone rispettava ed amava, però mi sento di attribuirgli il peso della tradizione del Risorgimento. So che Leone ha significato moltissimo nella storia del cattolicesimo organizzato. Per Leone quella storia iniziava molto prima che l'appello ai liberi e forti e quanto alla Costituzione repubblicana, di cui fu maestro, per Leone antifascismo e Resistenza significavano tutto tranne che un potere o, peggio ancora, un monopolio di parte. Leone non aveva difficoltà a sentirsi onorato di avere la tradizione della Resistenza degli Arrigo Boldrini, dei Giancarlo Pajetta, ma non ha mai avuto la viltà, colleghi della sinistra, di cancellare da questa storia né Randolfo Pacciardi né Edgardo Sogno. Ecco perché quel discorso su Crispi che aveva ascoltato a Napoli da ragazzo insieme a suo padre Mauro ne ha condizionato un momento altissimo si riflette una delle più degne tradizioni della nostra storia patria della quale credo che quest'Assemblea debba essere sempre riconoscente. Termina così la commemorazione della figura di Giovanni Leone in occasione del centesimo anniversario della nascita. Il Senato ha reso, in modo unanime, omaggio ad un eminente giurista, ad un uomo onesto, ad un grande Presidente della Repubblica. Il Senato non può - non è purtroppo nei nostri poteri - annullare le amarezze dell'ultima fase della sua Presidenza, ma può - e lo ha fatto oggi - rendergli l'onore dovuto con una sola voce.

Valori, UDC, SVP e Autonomie e Misto hanno avanzato la richiesta di procedere all'elezione di altri senatori Segretari. Su tale richiesta si è espresso il Consiglio di Presidenza. In base a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti i due senatori che essendo iscritti ai Gruppi richiedenti otterranno il maggior numero di voti, limitatamente ad un senatore per Gruppo. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Isenatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta. Dopo l'effettuazione della chiama, le urne resteranno aperte, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno. Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere alla chiama.

Grazie, *(IdV)*. Signor Presidente, ho preso la parola perché voglio leggere ai colleghi una lettera che ho ricevuto da una dipendente dell'Alitalia,

per denunciare che anche la 45a convocazione della Commissione di vigilanza RAI non ha eletto il Presidente e quindi non è stata insediata banchi della maggioranza).* Visto però che c'è stata partecipazione al voto, non si riesce a capire cosa osti a convocarla ad oltranza. Questo è l'unico modo per arrivare finalmente all'insediamento di questa Commissione, che è di rilevanza costituzionale.

Barelli, Bassoli, Bastico, Battaglia, Belisario, Benedetti Valentini,

in particolare dai lombardi, ma non solo. Alessandro Maggiolini nacque a Bareggio, un bel paese vicino al Ticino, a circa 20 chilometri da Milano. Tanti di noi

molto amato. *Spesso, però, in questo strano Paese le sue prese di posizione, le sue idee hanno suscitato polemiche, in particolare quando ha affrontato temi politicamente sensibili

«Cari bambini, tra una settimana è Natale, ma Babbo Natale non esiste; non è lui a portarvi i doni, ma papà e mamma rintronati dalla pubblicità. E non esiste neanche la Befana, che tra l'altro è pure brutta. Non piangete, non fate così. Gesù bambino, lui esiste, ma ha cose più serie da fare che andare in giro a portare i pacchi». pacchi». Questo era Maggiolini, e questo era il Maggiolini da noi molto amato. Molto più semplicemente, le sue idee erano così amate perché erano quelle della terra, della sua gente.

del non tenere nascoste alcune posizioni, che magari possono anche apparire scomode agli occhi dei più, ma che contribuiscono a determinare un pensiero più chiaro e più forte.

Colleghi, non possiamo affrontare in modo surrettizio, a partire da un richiamo all'ordine dei lavori, questioni di fondo che vanno disciplinate, a mio avviso, con altri strumenti.

ma il principale è quello che lo riguarda nel suo insieme e che ci consente in qualche modo di considerarlo una sorta di metafora dell'approccio a questi problemi che la maggioranza pratica e che temo intenda praticare nel seguito della legislatura. Dico che si tratta di una metafora e cercherò di spiegarlo articolando il mio pensiero su alcune delle norme più emblematiche, aventi - appunto - quasi carattere simbolico e metaforico di tale approccio.

È molto interessante riflettere sulla storia di questa norma e su come nella sua prima versione fosse stata presentata come una sorta di adempimento di un contratto stipulato con gli elettori; in cui, per l'appunto, la repressione cieca, irrazionale e spietata della mera situazione di clandestinità nel territorio dello Stato diventava uno dei punti fondamentali.

Era una delle bandiere del provvedimento e si è dichiarato che, con questa norma, si sarebbe fatto fronte al problema dell'immigrazione realizzando un effetto di formidabile deterrenza rispetto agli ingressi illegali nel territorio dello Stato. Non intendo fare la storia del dibattito su questa norma, né desidero sottolineare con eccessiva enfasi l'ingloriosa fine di quella norma nel momento in cui è andata a sbattere contro le indicazioni europee, dopo che erano state trascurate tutte le riflessioni da noi suggerite sulla palese incostituzionalità, oltre che sulla inciviltà e, mi sia consentito, anche sul carattere antiestetico di un provvedimento di questo genere. Sta di fatto che, per non perdere la faccia, il reato non è stato semplicemente cancellato, come sarebbe stato segno d'intelligenza politica e d'intelligenza in generale, perché di fronte agli errori la cosa più intelligente da fare è riconoscerli e passare avanti. Quel reato originariamente era un delitto punito con la pena fino a quattro anni e, addirittura, l'arresto obbligatorio in flagranza; tutti quanti tra noi hanno un minimo di dimestichezza con il funzionamento degli uffici giudiziari avevano facilmente pronosticato che quella norma avrebbe paralizzato in maniera pressoché irreversibile il funzionamento del sistema giudiziario. Ebbene, invece di limitarsi a cancellare questa norma e questo delitto, si è trasformato l'articolo e la fattispecie in una contravvenzione in una contravvenzione che è molto interessante per chi si diletta di mostri giuridici e in particolare per i teorici del diritto penale, i quali su questa norma possono esercitarsi a ritrovare in una unica singola concezione normativa una serie molteplice molteplice e variegata di contraddizioni con la Carta costituzionale, di profili di irrazionalità e, scendendo sul territorio che più interessa chi ha elaborato il provvedimento, di assoluta, radicale, sconfortante inutilità. tratta, infatti, di una contravvenzione non oblabile,punita con l'ammenda da 5000 a 10.000 euro, che darà naturalmente luogo ad un numero enorme di fascicoli processuali, che andranno a loro volta ad intasare uffici giudiziari che, se Dio vuole, non ne avevano proprio bisogno e che non produrrà alcun effetto dissuasivo.

8.000 euro? Se non fosse questione fin troppo seria il quadro complessivo in cui si iscrive questa norma, ci sarebbe davvero da farsi qualche qualche sana risata. Una cosa intelligente sarebbe semplicemente cancellarla, non già perché la norma così com'è produrrà danni diversi dal riempire gli armadi di qualche giudice di pace, ma perché sarebbe segno - ripeto - di intelligenza politica e un messaggio di resipiscenza rispetto ai modi di affrontare problemi seri, che non si possono affrontare con comportamenti e elaborazioni di norme che seri non sono affatto.

e si iscrive nel mosaico metaforico di cui parlavo e che cercherò di tratteggiare brevemente e terminando forse anche prima dell'esaurimento del tempo che mi è assegnato. Un'altra norma,

è quella dell'articolo 39, che prevede la possibilità di trattenere fino a 18 mesi un cittadino straniero ai fini dell'identificazione. Credo che noi per troppo tempo - e intendo soprattutto la nostra parte politica - abbiamo avuto la cattiva abitudine di tollerare le manipolazioni verbali che nascondono concetti gravi. Questi 18 mesi sono di galera. Sia ben chiaro! Il cittadino straniero non identificato, non già per sua resistenza, ma ad esempio perché non c'è collaborazione da parte dello Stato Stato dal quale lui abbia indicato di provenire o per le più varie ragioni dipendenti dall'inefficienza degli uffici pubblici o dallo stato patologico del soggetto che non è in grado di chiarire la sua posizione, può essere di chiarire la sua posizione, può essere trattenuto in quello che oggettivamente è un carcere, per un periodo di tempo - tanto per darvi un *in**put* della pratica degli uffici giudiziari - che equivale più o meno a quello che si trascorre in carcere per una tentata estorsione o per una tentata rapina: galera amministrativa. Nessuno tra noi si nasconde la necessità anche di intervenire spiacevoli ma indispensabili per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ivi inclusa una temporanea e il più possibile ridotta nel tempo

Ebbene, su tale aspetto si può discutere, e lo si potrebbe fare veramente se ve ne fosse la disponibilità. Purtroppo, su questi temi non solo non la registriamo, ma percepiamo, nel momento in cui offriamo una disponibilità al dialogo, un atteggiamento di chiusura una delle componenti ideologiche più gravi contenute in questo provvedimento bandiera, provvedimento metafora, provvedimento inutile e dannoso. *(**Commenti* Presidente mi autorizza, avrei piacere di proseguire. Vede Presidente, i dati statistici, che sicuramente chi ha prodotto queste norme conosce norme conosce (perché se non li conoscesse dovremmo davvero preoccuparci di un difetto di diligenza nella più delicata delle attività dei pubblici poteri, che è quella della produzione delle norme), ci informano di un dato altamente significativo: l'identificazione viene realizzata nei primi due mesi o, salvo casi rarissimi, non viene realizzata. Quindi, questa misura custodiale, questa galera amministrativa è inutile, dannosa, vessatoria e - non dimentichiamocelo - in un periodo in cui i tagli piombano come mannaie da tutte le parti, anche negli ambiti più delicati dell'esercizio dei poteri pubblici come la scuola, costosa, costosissima, perché questa gente in queste galere amministrative deve essere mantenuta dei costi che vengono fatte sono pressoché ridicole. Ulteriori enormi, inutili spese in situazioni in cui già sappiamo dall'analisi dei dati statistici che alla scadenza dei 18 mesi nulla sarà accaduto e si sarà semplicemente irrogata una costosa, non giurisdizionale, incivile misura detentiva. Metafora, abbiamo detto, della punizione virtuale e fantasiosa della clandestinità. Abbiamo detto di questa forma di punizione, molto meno virtuale, molto più reale, concretamente incidente sulla carne, sul sangue e - mi sia consentito - sulla pelle delle persone. E arriviamo all'articolo 44, veramente una chicca: la schedatura dei *clochard*, la schedatura dei barboni, dicendolo in italiano. Dalle rilevazioni statistiche, anche queste sicuramente note a chi ha elaborato questi provvedimenti, ma singolarmente ignorate, si tratta della categoria con livello di pericolosità sociale più basso in assoluto. I barboni sono non solo innocui, ma l'anello più debole di una catena sociale che, scendendo verso il basso, diventa sempre più dolorosamente vulnerabile in qualche modo il senso di colpa della nostra società. I sensi di colpa si possono affrontare in molti modi: o da uomini civili, cercando di rimuovere il problema e partendo dal presupposto che (se mi è consentito fare riferimento ad un concetto religioso) siamo tutti figli dello stesso Dio e non figli minori e disgraziati alcuni e altri che, per ragioni di censo o di fortuna, hanno diritto a maggiori privilegi, oppure semplicemente eliminando il problema, spazzando via come la polvere sotto il tappeto ciò che fastidiosamente ci ricorda la tragedia della disuguaglianza.

alcuni esponenti del centrodestra, chiacchierando nei corridoi, che questa schedatura in realtà serve per aiutare i barboni. Ottima cosa. Ma allora creiamo un registro di costoro presso il Ministero degli affari sociali e stabiliamo, nel momento in cui prevediamo una sorta di anagrafe dei barboni, anche una serie di conseguenze per loro positive dell'iscrizione in questo registro. Non ho visto conseguenze positive in questa norma. In realtà non vedo conseguenze di nessun tipo, tranne l'introduzione di una tecnologia sociale che è una tecnologia di puro controllo, anche qui metafora di una società del chiavistello. Vedete, la maggioranza si è data il nome di Popolo della Libertà, ma il quadro fosco e inquietante che viene da queste norme è quello di un partito della galera sociale.

galera sociale.

signora Presidente. Ove non fossi stato abbastanza chiaro, ripeto: metafora di una galera sociale. sociale. Cosa significa tutto questo e a cosa allude? Qui non si tratta di cattiveria o di bontà; ci può essere anche questo, ma riguarda le singole persone.

ronde. Ho qualche dubbio in più sul fatto che certi studi sulla psicologia dei gruppi siano noti a chi ha elaborato tale norma,

non parto dal presupposto, come pure potrebbe accadere, che in queste ronde si infiltrino deliberatamente dei violenti per poter sfogare le loro pulsioni in situazioni in cui credono di poter essere tutelati. Prescindo da questa ipotesi patologica - che pure potrà verificarsi e ipotizzo invece la situazione normale di un gruppo di normali cittadini che, esausti per la situazione di difficoltà sociale che in certe zone del territorio in cui abitano si è venuta a creare, pattugliano con il benestare degli

che costoro non gli stanno andando dietro non già perché sono onesti cittadini che pattugliano la loro città, ma perché sono soggetti uguali a quelli che hanno compiuto alcuni degli orribili atti di razzismo che abbiamo visto negli ultimi tempi? Che cosa ne sa lui? Scappa. Magari lo acchiappano e lui prova a difendersi, e se prova a difendersi costoro cercheranno di immobilizzarlo perchè, una volta che si innesca una colluttazione (chiunque vi si sia trovato lo sa), è molto facile cominciare, ma è molto difficile finire e soprattutto è molto difficile capire dove si andrà a finire. Vedete, un poliziotto o un carabiniere è addestrato a fare certe cose, è addestrato anche ad un uso misurato della violenza quando questa è assolutamente indispensabile. Io non faccio l'ingegnere, né il chirurgo e se mi chiedessero di fare un intervento chirurgico adesso ovviamente rifiuterei, perché potrei causare soltanto danni. Il lavoro del poliziotto o del carabiniere, il lavoro di chi per strada opera per garantire davvero la sicurezza è un lavoro difficile, che richiede professionalità, cosa che sembra ignorare chi ha redatto questa norma, ma che non ignorano quei tanti poliziotti, carabinieri e in generale appartenenti alle forze dell'ordine che, se andate ad interpellare adesso, sono terribilmente preoccupati per quello che può derivare dall'approvazione di una norma come questa. Presidente, non ho nessun problema: quando vengo interrotto mi fermo e aspetto che l'interruzione cessi. COLLI *(PdL)*.

il rischio di gravi danni. E non mi si venga a raccontare la storia dei nonni che vigilano davanti alle scuole, perché quelli già ci sono. Si tratta di un meccanismo del tutto diverso e, soprattutto, non si fa riferimento a quel pericolosissimo concetto di presidio del territorio che pare alludere ad un trasferimento delle potestà di polizia a gruppi di cittadini privi della competenza, dell'addestramento, dell'attitudine mentale - e prescindo dai profili morali - per esercitare il presidio del territorio, che è una delle prerogative ineludibili fondamentali dello Stato di diritto. Concluderò questa rassegna di norme, che - ripeto - ho estratto dal provvedimento per il loro particolare valore simbolico,

sia obbligatoria la custodia in carcere. Tutti sappiamo che la norma è ricalcata, o meglio è articolata sul precedente disposto del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che prevede l'obbligo della custodia cautelare in carcere, laddove esistano gravi indizi, per i reati di mafia e connessi.

e che implicheranno, ogni qual volta emergano i gravi indizi di colpevolezza, l'inevitabilità della custodia in carcere. Vorrei chiedere, e purtroppo non posso farlo perché non sono presenti in Aula, che cosa pensano di questa norma e della filosofia, dell'ideologia che c'è dietro di essa tutti gli avvocati penalisti appartenenti alle camere penali che, in passato, giustamente, hanno fatto battaglie il cui cuore, il cui nucleo era la tutela della libertà, che in questo provvedimento in modi

nefasti delitti che avvenivano nel nostro territorio. La Lega Nord da sempre si è battuta e si batte per questo problema. Ricordo che già nel 1995 iniziavamo a tenere, in tempi non sospetti, le prime riunioni in cui parlavamo dell'aumento indiscriminato della microcriminalità che derivava dall'ingresso degli extracomunitari nel nostro territorio. La Lega Nord - dobbiamo riconoscerlo - ha sempre spinto in questo senso, perché fin da subito, in anticipo sui tempi, abbiamo capito che dal punto di vista normativo eravamo sicuramente impreparati a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione, di questa forzata globalizzazione dei popoli. Sono passati i periodi in cui si è scherzato sul problema sicurezza. E si è scherzato parecchio, si è scherzato parecchio, cari amici della sinistra, perché emanare due decreti-legge sulla sicurezza e poi non avere né la forza, né il coraggio di convertirli in leggi significa scherzare sulla pelle dei cittadini. Fare un provvedimento come quello sull'indulto, che sicuramente il senatore Carofiglio avrà approvato, significa scherzare sulla sicurezza, sulla pelle di tutti quanti i cittadini italiani. L'Italia tutta ha vissuto recentemente un momento storico di notevole grigiore: l'invasione dei rom e degli extracomunitari in genere, da alcuni dipinti come una risorsa per noi e per il nostro Paese, in nome di quel falso buonismo di sinistra che vuole il nostro territorio, l'Italia, un porto di mare in cui facciamo entrare tutti, senza pensare a quello che succede dopo a queste persone. Troppo spesso, queste persone non hanno una casa, troppo spesso queste persone non hanno un lavoro, troppo spesso queste persone vengono utilizzate nei circuiti

I numeri, signora Presidente, ci danno ragione: ci sono carceri in Italia in cui abbiamo il 70-80 per cento di cittadini extracomunitari, e questo sicuramente ci fa rabbrividire, ma ci fa anche pensare che abbiamo ragione nel dire quello che diciamo.

limiti ai flussi migratori, regole certe per fronteggiare l'illegalità diffusa, la criminalità organizzata, per garantire la sicurezza urbana. Questo volevano i cittadini, questo hanno voluto i nostri elettori che, come sapete, cari amici della sinistra, sono tanti.

Abbiamo zone in Italia nelle quali non è più possibile parlare di integrazione, quando si determinano situazioni come quelle di alcuni paesi o di alcune province del Nord, dove si raggiungono concentrazioni di cittadini

Credo che il Ministero sia sicuramente sulla strada giusta perché li sta colpendo su quello che hanno più a cuore: il sequestro dei loro beni, quindi il denaro. Adesso parliamo di un argomento sicuramente delicato (ne ho sentito parlare anche quest'oggi in Aula diverse volte): parliamo della possibilità data ai cittadini e ai sindaci di poter aiutare le forze dell'ordine nel controllo del territorio. Questo, secondo me, è senso civico, cari amici di sinistra che tanto avete parlato di questo provvedimento, che, tra altro, è l'articolo 46 del disegno di legge n. 733. Questo è senso civico

il rispetto per lei, Presidente - di quello che succedeva nel territorio, ma vi preoccupavate di quello che facevamo noi. Forse eravamo una deriva istituzionale? No, non credo.

eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio». In queste poche righe credo non si nasconda nessuna deriva istituzionale. Non lo credo Aumenterà sicuramente - come ho detto prima e ho ribadito diverse volte - il senso civico e di comunità. Se le regole vengono rispettate - credo - ne abbiamo tutti da guadagnare, anche gli extracomunitari extracomunitari che con l'accordo di integrazione potranno dimostrare di saper convivere civilmente nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, magari anche rispettando i nostri usi, costumi e tradizioni. Credo che questa sia la strada giusta.

di indumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, il famoso *burqa*, tanto per capirsi. Credo che se non si ha nulla da temere non si deve nascondere la propria faccia. E non si dica, cari colleghi, che queste persone lo fanno perché sono le loro tradizioni, usi e costumi perché, oltre ad una questione di sicurezza, è anche una questione di rispetto. Infatti, quando noi andiamo all'estero

Dietro ad uno di questi indumenti potrebbe tranquillamente nascondersi chiunque, un delinquente o un terrorista, come è successo a Londra negli attentati del triste luglio 2005 che tutti quanti ricordiamo. Mi sento di Mi sento di rivolgere in questa sede un sentito e doveroso ringraziamento agli amici del Popolo della Libertà perché ci hanno seguiti sulla strada del rafforzamento della legalità, condividendo e sottoscrivendo lo sforzo del nostro movimento, la Lega Nord, che con questo disegno di legge farà sì che i cittadini recuperino quella fiducia e quella tranquillità che negli ultimi anni era andata perduta. Agli amici di sinistra vorrei invece rivolgere un invito sentito e sincero ad abbandonare la strada sterile e demagogica del dover essere a tutti costi sempre e contro tutti. Vi rendete conto, cari amici di sinistra, che siete contro la sicurezza dei vostri e dei nostri cittadini? I cittadini sono di tutti. I cittadini, una volta finite le elezioni, non hanno più colore politico. Oltre che contro i cittadini siete contro i vostri stessi sindaci:

che hanno posto in essere il controllo del territorio e stanno chiedendo a gran voce maggiore sicurezza nei loro territori. Se non volete ascoltare noi, almeno ascoltate i sindaci che sono vostra espressione politica. Abbandonate, cari amici, quel sinistro atteggiamento di negatività. La sicurezza, dicevo prima, non è di destra o di sinistra; anche i cittadini che a suo tempo vi votavano se ne sono accorti, e i risultati li avete visti.

ai familiari di quella povera coppia di coniugi che sono stati trucidati nell'agosto dello scorso anno. Ecco, credo sia finito il tempo della sterile demagogia; si pensi realmente a fare le cose concrete. Con il disegno di legge che stiamo approvando sicuramente faremo qualcosa di concreto. colleghi. il provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica è la risposta alle esigenze avvertite dalla società civile, quotidianamente sempre più colpita da atti di criminalità di varia natura, in special modo tra gli strati sociali più poveri. Il disegno di legge n. 733 assorbe infatti altri disegni di legge presentati da altri schieramenti sul medesimo tema della sicurezza. In tutti credo vi sia l'obiettivo di aggiornare il nostro sistema giudiziario alle nuove esigenze di ordine pubblico. Infatti, il sistema così com'è non funziona. È positivo quindi che le nuove norme volte a contrastare reati legati alla criminalità organizzata e ad apprestare strumenti di tutela per gli anziani, gli handicappati ed i minori guardino anche a crimini secondari, come l'imbrattamento degli immobili (con norme che ne migliorano il contrasto), e prevedano misure per il rafforzamento delle sanzioni agli automobilisti ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con l'obbligatorietà della pena accessoria della revoca della patente di guida. tutte norme che vanno incontro ad una necessità reale ed obiettiva: quella della legalità e della percezione della legalità da parte dei cittadini italiani, ma anche di coloro i quali transitano nel nostro Paese, sia come turisti, sia come soggetti in cerca di un onesto lavoro. Provengo da una Regione, la Sicilia, dove l'attenzione a uno di questi temi che stiamo affrontando, quello dell'immigrazione, è molto forte. Sappiamo tutti che le nostre coste contano ormai troppi sbarchi di clandestini e che i CIE (Centri di identificazione e di espulsione) in Italia, soprattutto nel periodo estivo, sono al limite della loro capacità di accoglienza. A questo occorre aggiungere l'oggettiva difficoltà da parte delle forze dell'ordine di identificare i soggetti, alcuni dei quali arrivano anche ad ustionarsi i polpastrelli per evitare il riconoscimento Molti di essi sono persone già espulse da nostro Paese e che tentano nuovamente la strada disperata dello sbarco sulle nostre coste, mettendo a repentaglio, come sappiamo e come abbiamo visto tante volte, anche la loro stessa vita. Dobbiamo poi considerare anche coloro i quali riescono ad eludere i nostri sistemi di sorveglianza e che sono destinati quasi sempre ad una vita misera, fatta di sfruttamenti, accattonaggio, in buona sostanza di condizioni di vita non degne di un Paese come l'Italia, che li ospita. Ma non dobbiamo pensare che l'immigrazione illegale provenga soltanto dal mare. Le cronache quotidiane dei giornali e le televisioni ci dicono che le popolazioni dei Paesi dell'Europa dell'Est (come la Romania, la Bulgaria, l'Albania) hanno colonizzato le città italiane. Questo è un mercato del lavoro in cui persino i nostri cittadini faticano ad andare avanti e a trovare spazio. La scontata evoluzione nella vita clandestina di questi soggetti con poche risorse e alloggi di fortuna è purtroppo quasi sempre negli affari illegali, nei mille episodi che riempiono la cronaca di tutti i giorni, nell'alcol, nel baratro dei vari *racket* che li sfruttano e, soprattutto, in una vita fatta di non integrazione. Tale stato di cose penalizza tutto: penalizza i cittadini italiani, sempre più impauriti e esasperati da una delinquenza anche spicciola, ma penalizza anche quelle fasce di immigrati che si sono perfettamente integrati, che lavorano, che sono utili al Paese e che cercano di avere una vita decorosa ed onesta. Questi svolgono anche dei lavori che ormai molti italiani non vogliono più fare: nelle famiglie come badanti, nelle fabbriche come operai, nelle realtà agricole come braccianti. In questa situazione abbiamo due grosse responsabilità: la prima nei confronti dei nostri cittadini e di coloro che vivono onestamente in Italia, con il diritto che hanno e che abbiamo tutti alla sicurezza; la seconda nei confronti degli stessi clandestini, perché uno Stato democratico come il nostro deve poter garantire a tutti accoglienza, cure e assistenza nel rispetto dei diritti umani ma anche, e soprattutto, delle leggi vigenti. Per questo motivo ritengo giusto frenare l'ingresso indiscriminato di persone che vengono in Italia in cerca di fortuna, in quanto il nostro sistema di accoglienza ormai è saturo e non consente più un'incontrollata affluenza in massa di forza lavoro. La comune coscienza democratica deve fare i conti con questa realtà (soprattutto con questa realtà), individuare il problema e porvi di conseguenza rimedio. Proprio in questa direzione si muove l'articolo 9 Esso, infatti, introduce nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, con annesse sanzioni obbligatorie. La *ratio* del provvedimento è evidentemente quella di innalzare il livello di prevenzione per questo reato. Anche altri Paesi europei (come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania) hanno nel proprio ordinamento giudiziario questa norma e sono Paesi che prima di noi hanno dovuto affrontare questi problemi. Oggi da noi l'immigrazione clandestina è un reato punibile solo a livello amministrativo. Di fatto, vi è una non punibilità del reato stesso che ha solo alimentato le speranze di quanti affrontano viaggi disperati in mare o con mezzi di fortuna, con il miraggio di condizioni di vita migliori. Di quanti espatriano perché nel proprio Paese non hanno futuro e mirano a migliorare le condizioni di vita personali e delle proprie famiglie ormai è pieno il nostro Paese. A tutti questi noi non possiamo, non dobbiamo, offrire illusioni e alimentare speranze ingiustificate.

Proprio per questo motivo si è provveduto a identificare e colpire chi specula su queste situazioni. Pensiamo, ad esempio, alla modifica della disciplina del reato di agevolazione nella permanenza di stranieri irregolari oppure al reato di favoreggiamento di clandestinità. La mancanza di punibilità, infatti, non alimenta soltanto speranze, ma anche e forse soprattutto il proliferare di affari lucrosi di quanti vivono e speculano sulla disperazione altrui. Le organizzazioni criminali transnazionali hanno trovato facile terreno nel nostro Paese in questo settore. È un'industria della malavita che organizza di tutto (dalle tratte dei clandestini, ai matrimoni a distanza, a consegne di tutti i generi) e che sposta capitali di dubbia provenienza grazie a numerosi buchi della nostra legislazione, utilizzando anche le tecnologie informatiche più avanzate. Proprio sulle leggi vigenti bisogna porre l'attenzione. Abbiamo detto che queste non funzionano così come dovrebbero: lo dicono i fatti e lo dicono a gran voce i cittadini, che sono esausti, preoccupati e terrorizzati di vivere in una situazione di non sicurezza o di poca sicurezza.

proverò a sintetizzare nel mio intervento tre aspetti, due dei quali apparentemente formali,

parlare già la settimana scorsa sui provvedimenti che riguardavano pure la sicurezza. Parte del mio intervento sarà poi dedicata al merito, cioè all'efficacia alla capacità di queste misure di conseguire almeno gli obiettivi che il provvedimento si prefigge. Ancora una volta, anche in questa circostanza, sono preoccupato per la certezza che ho che alcune delle norme contenute in questo disegno di legge, soprattutto alcune delle norme introdotte dagli emendamenti del lavoro delle Commissioni confliggano in maniera significativa con le disposizioni della Costituzione. Questa mattina i colleghi, nelle eccezioni di costituzionalità, hanno avuto modo di dimostrare che, ad esempio, nell'uso che si fa dell'istituto del matrimonio, che è di garanzia e previsione costituzionale, e dell'intreccio tra questo istituto e la cittadinanza

la nostra Carta costituzionale costituisce un patrimonio che, a mio avviso, va difeso. Almeno in quella, dobbiamo riconoscerci e ritenerla come un patrimonio che tiene insieme le diverse opinioni e i diversi modi di vedere le tante questioni, le tante sofferenze e i tanti problemi del nostro Paese. Sono poi preoccupato perché molti istituti introdotti hanno una complessità di gestione, la annunciano. Mi meraviglia che non vi sia, né vi sia stata un'analisi della gestione dei provvedimenti, sia di quelli di competenza delle forze dell'ordine e di polizia, sia da parte della magistratura.

e a produrre un effetto rassicurante che non a caricarsi della soluzione del problema, introduciamo istituti più complessi di quelli che fin qui l'ordinamento giudiziario ha avuto modo di gestire,

che non dico sovvertono, ma rendono ancora più complesso l'ordinamento giudiziario e la gestione della giustizia nel nostro Paese. Entrambi i temi (l'ordinamento costituzionale e l'ordinamento giudiziario) mi premono, oltre che per le ragioni culturali e politiche, per gli aspetti che attengono alle fondamenta della democrazia del nostro Paese

di certezza e di chiarezza negli istituti che dovrebbero affrontare il tema generale della legalità nel nostro Paese, abbiamo

smentire che una norma e la severità dei provvedimenti che si accompagnano ad una norma possano avere una funzione deterrente. Se però immaginassimo che esclusivamente nella severità delle norme possa sintetizzarsi la soluzione al problema commetteremmo un gravissimo errore

che più attività debbono concorrere a rimuovere un problema. Questo provvedimento, i provvedimenti di severità così definiti hanno un senso se sono preceduti da forti azioni e da forti provvedimenti che attengono, in primo luogo, alle politiche sociali.

neppure dopo i provvedimenti che erano stati annunciati come decisivi, definitivi, risolutivi della questione. Anzi, noi registriamo un fenomeno addirittura contrario, cioè un incremento:

risolutiva e definitiva dei problemi della criminalità e dovessimo invece registrare, da qui a qualche tempo, che nessuno degli effetti sperati si è realizzato, saremmo in presenza di uno Stato che ha caricato un'aspettativa fortissima sull'ultima delle sue spiagge possibili, vale a dire la legislazione speciale

a svolgere compiti di presidio del territorio, espressione non solo generica, ma che introduce una categoria di attività che non si tratta? Forse è la sicurezza integrata? Su quella strada, però, il nostro Paese si era già incamminato ed aveva in qualche modo già attivato forme e procedure di integrazione tra le forze dell'ordine: molti sindaci avevano disposto protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, adeguando e mettendo a disposizione i vigili urbani.

dell'attività di ordine pubblico associazioni di cittadini che si mettono in campo per un senso civico, per un dovere civico. Inoltre, quel dovere civico della segnalazione può essere esercitato anche singolarmente e non è l'azione collettiva che ne determina la possibilità. Concludo, signor Presidente, dicendo che in questo caso, come per quanto riguarda le forze dell'ordine, leggo un implicito giudizio di inadeguatezza di coloro che, invece, sono predisposti ai compiti di sicurezza pubblica nel nostro Paese.

che, invece, dobbiamo affrontare: se la sicurezza è al centro delle questioni di questo Paese, la risposta non può essere in queste soluzioni, ma sta al centro della questione, cioè nel rafforzamento coloro che sono naturalmente predisposti a tutelare l'ordine pubblico del nostro Paese. La risposta, dunque, è semplice: più poliziotti, più carabinieri, più forze dell'ordine, più strumenti dedicati a loro per la prevenzione e per la repressione. Tuttavia, non si può da un lato annunciare il tema, propagandarlo, farlo anche consensi elettorali e poi registrare che nelle manovre finanziarie i fondi predisposti a chi quotidianamente con sacrificio si occupa della nostra sicurezza

sia un reato nel reato. Noi non apparteniamo a quella schiera; però non vogliamo neanche appartenere alla schiera di chi ritiene

devo dire che sono piuttosto sconcertato, forse perché sono un uomo prestato alla politica e un tecnico che per 45 anni si è occupato di lotta alla criminalità,

elaborato questo disegno di legge, quando suggerivamo - e lo abbiamo fatto a gran voce - che il modo migliore per combattere la criminalità organizzata, secondo un'opinione che si sta diffondendo in tutti i Paesi occidentali, è agire invertendo l'onere della prova. Abbiamo sempre detto che la corruzione, l'evasione fiscale e la criminalità organizzata si combattono proprio invertendo

siano fatti determinanti e quasi esclusivi per scoraggiare la criminalità. E allora non si rimane solo sorpresi, ma

una pena fino a quattro anni di reclusione per il reato di immigrazione clandestina si sarebbero scoraggiati gli arrivi. Mi sembra un *déjà vu*, come del resto è stato anche con la legge Bossi-Fini.

come procuratore della Repubblica di Milano, di essere interpellato e visitato ufficialmente dal Capo dell'ufficio immigrazione degli Stati Uniti d'America.

del senatore Carofiglio, il quale, essendo in Parlamento, ha diritto di dire la sua anche se può essere cosa non piacevole e non grata alla maggioranza

soprattutto fornendo aiuti e impedendo che questi poveri disgraziati finiscano vittime di quelli che sono veramente gli autentici colpevoli, coloro che pongono in essere una sorta di tratta degli esseri umani. Noi, invece, abbiamo seguito una strada completamente diversa. Ebbene, ancora mi sono trovato a dover affrontare la cosiddetta criminalità diffusa. Mi dispiace

Comunque, senatore Ferrara, gradirei non essere interrotto. Non ho mai interrotto nessuno di voi né mi sono spostato sui banchi per dire improperi. A questo punto, educatamente, cerchiamo di discutere di questioni serie con grande serietà.

in cui si diceva «Vietato l'ingresso ai cani e ai meridionali». Eppure i meridionali hanno prodotto il *boom* sono stati loro, quelle braccia a basso costo che venivano dal Sud che hanno reso possibile il *boom* economico, così come adesso molta della ricchezza prodotta al Nord nelle Regioni della Lega è stata portata proprio dagli immigrati,

di invasione dei rom, dimenticando che la maggior parte di loro è nata in Italia.

Quindi, abbiamo risolto i problemi di sicurezza o li abbiamo aggravati? Per quanto mi risulta, i rom ci sono dall'anno 1000 dopo Cristo e sono stati sempre nomadi.

com'è stato già fatto notare, allora gli altri saranno spinti, se non si adottano contemporaneamente dei provvedimenti sociali, a diventare delinquenti.

aiuto sociale. Allo stesso modo, per la sicurezza, sarebbe stato molto meglio togliere alla Polizia una serie d'incombenze amministrative, quali il rinnovo dei permessi di soggiorno e affidarle ai Comuni, che conoscono meglio la situazione e sanno bene quel che devono fare.

Ebbene, l'anno successivo la criminalità è diminuita del 30 per cento. Sono queste le esperienze serie di cui bisogna tenere conto e non le chiacchiere che si fanno ad

ragionando su un disegno di legge che è completamente diverso da com'era stato presentato inizialmente e che è stato cambiato nel corso della discussione, anche con prove di buona volontà da parte di tutti, ma che in effetti viene discusso in queste condizioni Non credo si fornisca un buon servizio alla collettività in questo modo. Tra l'altro, discutiamo di un disegno di legge che fa parte del cosiddetto pacchetto sicurezza e che contiene norme eterogenee: eterogenee: norme in materia di immigrazione, di controllo sociale, di contrasto al crimine organizzato, di aggravamenti di reati contro la persona, contro il patrimonio, il decoro urbano, la circolazione stradale e anche interventi sul piano procedurale. Sono ormai disegni di legge o decreti‑legge a cui ci stiamo abituando e che sono una sorta di *omnibus*, per cui in un quadro già abbastanza complesso e difficile del nostro ordinamento giuridico, in cui si dovrebbe semplificare, andiamo a infilare una serie di tasselli che continuano a stravolgere complessivamente le norme sia sostanziali sia procedurali, con una distonia tra varie norme di cui ci accorgeremo poi nell'applicazione concreta e di cui pagheremo gravemente il prezzo. Si tratta quindi di un provvedimento complesso, di difficile lettura, che in parte riprende proposte contenute nel pacchetto sicurezza del governo Prodi, che sono condivisibili sempre che non siano state stravolte attraverso interventi aggiuntivi, con finalità forse anche buone ma che finiscono per vanificarne l'efficacia dissuasiva.

già forte disagio sociale, con la difficoltà - come diceva giustamente la senatrice Magistrelli - di pensare a questi bambini che verranno tolti alle famiglie e che dovranno pure essere affidati a qualcuno. Mi pare che questo aspetto del problema non sia stato minimamente approfondito. Vi sono poi altre disposizioni introdotte durante i lavori delle Commissioni riunite e mi riferisco in particolare ad alcune proposte di carattere costruttivo del Partito Democratico che sono state accolte dalla maggioranza, in particolare in materia di criminalità organizzata, di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, di tutela penale rafforzata nei confronti di soggetti vulnerabili, in particolare donne e minori, per alcuni aspetti e non per altri. È evidente quindi che l'opposizione e in particolare il Partito Democratico sosterrà queste norme anche in Aula. Mi sia consentito dire, però, che si tratta delle uniche norme che rispondono alla strategia di una politica tesa effettivamente alla sicurezza ed al contrasto dell'illegalità nel rispetto dei diritti umani, del diritto anti-discriminatorio, di principi costituzionali, di quelle norme comunitarie e di diritto internazionale vincolanti per l'Italia e in quanto tali costituzionalmente garantite. Altre norme appaiono invece decisamente improponibili, perché inutilmente lesive di diritti garantiti, discriminatorie e tali da allontanare il nostro Paese da principi costituzionali e da atteggiamenti propri di una società civile. In realtà, si sta svolgendo una pressione sempre più forte sul sistema costituzionale che finisce col rivolgersi pesantemente non solo a quella seconda parte della Costituzione, rispetto alla quale tutti forse vorremmo dei cambiamenti, ma soprattutto rispetto alla prima parte che contiene l'esposizione dei diritti. Viene posto così in discussione non solo il principio di uguaglianza ma tutto il quadro dei diritti. diritti. Ad una prospettiva di questo genere dovremmo opporci tutti trasversalmente perché credo che la tutela dei diritti umani, dei diritti riconosciuti universalmente, dovrebbe essere garantita a tutti. Ma questo non avviene e probabilmente perché si sta consolidando un'abitudine culturale, una sorta di assuefazione all'idea di una comunità chiusa, che coltiva - come è stato autorevolmente detto - distanza e ostilità, che alimenta il conflitto tra i gruppi sociali contigui, che giustifica le guerre tra poveri. Così finiscono con alzarsi barriere e si viene a predicare una tolleranza che si risolve in una accettazione dell'altro, del cittadino straniero considerato come un diverso, perché prevalentemente le norme sono dirette dirette a frenare l'immigrazione, alla sola condizione che questo cittadino straniero, quello diverso, faccia ciò che serve ai cittadini italiani, quello che i cittadini italiani non vogliono fare, alle condizioni quindi che noi imponiamo. Ma, esaurita questa funzione, possibilmente il diverso deve sparire per liberaci - come sempre ed autorevolmente è stato detto - da ogni inquietudine umana e sociale. Naturalmente a tale prospettiva il Partito Democratico si sta fortemente opponendo perché non solo è miope, ma manca di una qualsiasi visione strategica del problema della sicurezza e dell'immigrazione. E questo finisce con dare vita a norme che, forse non volute nemmeno da coloro che le hanno proposte, non risolvono ma anzi aggravano i problemi della sicurezza e della immigrazione irregolare, spingendo tra l'altro gli immigrati clandestini a cercare appoggio e protezione nella criminalità organizzata, proprio quella che tutti vorremmo congiuntamente combattere. Vorrei riprendere parole pronunziate da un esponente della maggioranza, universalmente apprezzato, il senatore Pisanu, che è stato Ministro dell'interno e che autorevolmente oggi è Presidente della Commissione antimafia. Se non erro nell'anno 2002 Pisanu così recitava: accorda assistenza umanitaria in base alle regole internazionali a tutti coloro che fuggono da carestie e guerre. Ma contrasta l'immigrazione irregolare, avendo l'obiettivo di favorire quella regolare». Gli immigrati clandestini, diventano un problema perché «inevitabilmente finiscono in mano ad affaristi o al crimine organizzato che li buttano sul mercato nero, se non addirittura nella prostituzione o nella manovalanza criminale». Ebbene, non c'è dubbio che le organizzazioni criminali possano trovare fra i disperati dell'immigrazione clandestina un terreno di reclutamento favorevole che queste organizzazioni, possano appaltare segmenti delle loro attività, le più sporche e rischiose, legate al controllo del territorio come lo spaccio e la prostituzione ad immigrati irregolari, col duplice vantaggio di sviare l'attenzione e di avere un esercito di manovalanza ricattabile e pronto a tutto. Eppure un percorso ad ostacoli per divenire cittadini regolari e tutti gli ostacoli posti per scoraggiare l'immigrazione e per punire gli immigrati finiranno col produrre - anche e forse senza che chi lo ha proposto lo abbia voluto - questi effetti. Parto dal testo emendato del disegno di legge, che introduce come contravvenzione punita con l'ammenda il reato di immigrazione irregolare, con un meccanismo che ignora le vittime di tratta e comunque i titolari dì un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Questo meccanismo non è conforme né ai principi costituzionali di legalità della pena, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, né a quelli di presunzione di innocenza, di eguaglianza di fronte alla legge e di effettività del diritto di difesa. Un collega della maggioranza si meravigliava di come potesse essere leso il diritto di difesa in questo caso: impedendo ad una persona di potersi difendere di fronte al giudice di pace, che è pur sempre un giudice e quindi ha diritto di avere il suo imputato. Sottrargli, in questo caso, il controllo sul visto significa creare una disparità di trattamento tra persone. Si finisce con questa ed altre disposizioni a dare vita ad un diritto speciale, fondato su una sostanziale sospensione di diritti e garanzie fondamentali che riguarda le persone. Così per lo straniero si finisce col costruire un diritto che lo discrimina e punisce in quanto tale, anche per comportamenti per i quali la sanzione penale è chiaramente impropria e sproporzionata, come nel caso dell'immigrazione irregolare, ovvero è ingiustificatamente diversa da quella prevista per altri soggetti che commettono lo stesso reato. Cito per tutte l'aggravante di pena per la semplice condizione di clandestino introdotta con il decreto-legge sicurezza del 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, In questo modo si continua a sovraccaricare di compiti inutili il sistema investigativo e giudiziario, a danno della sicurezza dei cittadini, mentre l'unica risposta seria all'immigrazione irregolare è costituita dall'espulsione. Ed è, invece, sotto questo profilo che servono strumenti e risorse che, nel rispetto dei diritti umani e sulla base di accordi con i Paesi di provenienza per un rimpatrio assistito (come proposto dal PD) rendano effettiva tale misura amministrativa, dando davvero impulso ad una strategia di contrasto all'immigrazione irregolare.

ulteriori disposizioni del disegno di legge che introducono il cosiddetto permesso di soggiorno a punti per i cittadini stranieri; estendono il periodo di possibile trattenimento sotto forma di detenzione amministrativa nei centri di identificazione, se vi sono difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero nell'acquisizione dei documenti per il viaggio (con una irragionevole e ingiustificata

subordinano il diritto al riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo al previo superamento di un test di lingua italiana; impediscono la celebrazione del matrimonio in Italia per gli stranieri che non esibiscano un documento attestante la regolarità del soggiorno (in violazione degli Una particolare attenzione poi deve essere rivolta al rimpatrio assistito dei minori comunitari, che si prostituiscono e quindi sono vittime di cui va invece favorita l'integrazione e la tutela. Proprio per i minori, di cui vanno affermati i diritti, viene recepito un trattamento deteriore e in contrasto con la direttiva n. 38 del 2004, già recepita con il decreto legislativo n. 30 che prevede che i cittadini comunitari possono essere allontanati solo per ragioni di pubblica sicurezza e di pericolosità sociale e per i minori in circostanze eccezionali. Non è una norma singola, perché, per quanto riguarda il rimpatrio assistito dei minori, qui si parla dei comunitari, mentre in un disegno di legge del Governo che riguarda la prostituzione si parla di ridurre drasticamente il sistema del rimpatrio semplificandolo: quindi, aggiungendo anche in questo caso qualcosa che preoccupa rispetto a coloro che spesso sono vittime del traffico di esseri umani. Altrettanto preoccupanti sono le norme inserite dalla maggioranza che riguardano il controllo sociale in senso lato, prevedendo il presidio del territorio da parte delle ronde. Vorrei dire che in questo caso erroneamente si dice che non ci sono poteri da parte dei privati di intervenire ad assistere la polizia giudiziaria nei suoi compiti istituzionali; basti pensare che per alcune fattispecie è obbligatorio nel nostro ordinamento denunziare e che il cittadino italiano può addirittura procedere in alcuni casi, quando l'arresto è obbligatorio, all'arresto facoltativo. Non vedo quindi perché si debbano aggiungere compiti rispetto a quelli che sono istituzionalmente attribuiti alla Polizia e che uno Stato deve garantire e che, secondo me, non solo per il rispetto della Costituzione ma per il rispetto di se stesso, deve avere la volontà ferma di garantire. Quindi, a parte l'inammissibilità di alcune scelte contrarie a principi costituzionali riguardanti l'uguaglianza e la stessa dignità delle persone, siamo in realtà di fronte a norme che possono far crescere inefficienza, generare irregolarità e perfino produrre contrasti. Già è stato detto molto su quello che potrebbe succedere con le ronde formate da cittadini, non attrezzati, nemmeno mentalmente e professionalmente, a svolgere il lavoro delle forze dell'ordine. In questo modo molto lavoro, spesso inutile, attende non solo le forze di polizia e la magistratura, ma anche la Corte costituzionale

Sia per l'ISTAT che per il *dossier* Caritas, la popolazione immigrata è aumentata di diverse centinaia di migliaia e ciò è avvenuto sia nel 2007 sia, come ricordava il senatore Chiurazzi, nel 2008, senza regolarizzazioni e quote aggiuntive e in un periodo segnato, tra l'altro, da un andamento economico negativo. Nella presentazione del *dossier* Caritas (quindi ormai il Parlamento è a rimorchio di quanto associazioni di vario genere, in questo caso un'associazione cattolica, pongono in evidenza), Franco Pittau sottolinea: "Questo radicamento, così forte anche in una congiuntura poco favorevole, richiama l'attenzione sulle parole che noi solitamente utilizziamo ("straniero" e "extracomunitario") e porta a concludere che le stesse iniziano ad apparire desuete

ai lavori parlamentari. Ritengo però opportuno sottolineare come, ancora una volta, siano le associazioni ad andare

che insista sulla maggiore convenienza delle vie legali dell'immigrazione e sulla collaborazione delle associazioni degli immigrati, anche perché prevenire costa molto meno che reprimere e i fondi a disposizione sono limitati. La situazione attuale è una palestra che aiuta a prepararsi al futuro, in cui italiani e immigrati sono chiamati a convivere. Forse varrebbe la pena di riflettere su questo e mi auguro che la maggioranza lo faccia, ritirando quelle norme inefficaci per la sicurezza e inutilmente lesive di diritti. Vorrei poi soffermarmi su due punti. Nel *dossier* Caritas si parla del tasso di attività dei cittadini stranieri, che

Eppure il grave sfruttamento del lavoro rappresenta oggi una delle più preoccupanti forme che assume il neoschiavismo; quel dominio dell'uomo sull'uomo che priva la persona della libertà, dell'autodeterminazione e della dignità. concerne le ronde, oltre ai profili di costituzionalità e all'inquietudine che la proposta fa nascere, vorrei chiedere seriamente: davvero pensiamo di doverci difendere solo all'esterno e con tutti i mezzi ( legittimi o meno) e non nelle mura domestiche italiane?

e che, contrariamente a quanto si dice, non sono in discussione alla Camera ? Lì si sta trattando la materia dello *stalking* ma, sicuramente, non di tutela delle vittime per quanto riguarda maltrattamenti in famiglia e l'incidente probatorio protetto. Su questa base, signora Presidente, l'invito che noi dobbiamo fare è per una riflessione approfondita rispetto a quella, molto superficiale, che è stata fatta (perché non si può riflettere in una notte) e per trovare un punto di incontro per quella tutela dei diritti umani che, come dicevo inizialmente, è una tutela trasversale.

a fare intendere che io sarei un bambino capriccioso. Per la verità, le battaglie da lei condotte in tutti questi anni mi hanno insegnato che, a volte, si conducono battaglie anche per asserire principi che non tutti, probabilmente, possono individuare subito.

era il mio intendimento, ma il divieto che qualcuno voleva porre nei confronti della mia voglia di partecipazione è un fatto gravissimo e solo quando ho avuto la certezza di poter partecipare - per rispetto verso i colleghi che là dentro rappresentano il Senato e me in modo degno - ho preferito uscire.

perché il centrosinistra - come abbiamo sentito in alcuni interventi svolti oggi - è inadeguato e ideologicamente impreparato ad affrontare tali tematiche.

che gli sbarchi clandestini non solo non sono restati quelli che erano, ma sono aumentati del 60 per cento

2008). Evidentemente, non godono della stessa pubblicità che avevano durante il Governo Prodi, ma questo è un dato di grande difficoltà, rispetto agli annunci delle politiche di contenimento.

e sbattuto in galera. Ma l'idea che da delitto sia diventato reato contravvenzionale con la previsione di un'ammenda (si immagina quindi che il clandestino sbarchi con la tessera del bancomat)

non solo di condivisione, ma di costruzione e di proposta di questi articoli. Restano non solo i punti critici che sono stati rilevati, ma resiste poi un punto di vista politico e culturale sul quale una differenza

In questi giorni è stata pubblicata la 18a diciottesima edizione del *dossier* statistico Caritas Migrantes, un osservatorio mai confutato e degno di

nel 2007 è stato di 3,74 miliardi di euro, contro un miliardo ristornato in termini di servizi; il contributo alla formazione del PIL, secondo la stima di Unioncamere, è del 9 (nel Veneto nel 2000 vi erano 20.000 imprese straniere, che utilizzavano lavoratori stranieri; oggi sono 40.000, sono

le mani nelle tasche dei cittadini, dovrebbero specificare «nelle tasche dei cittadini italiani», non di quelli stranieri, ma regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.

alla criminalità; vi è il tentativo di parificare molto spesso l'equazione, che ripeto ancora una volta, delinquenza-sicurezza-immigrazione.

di costruire un recinto più confortevole alla propria esistenza e alla propria presenza sul territorio, si inseriscono norme discriminatorie che nulla hanno a che vedere con la sicurezza. A questo

voluto non sprecare un'occasione importante su un tema così delicato, lasciando fuori le questioni che nulla c'entravano e concentrandoci davvero sulle emergenze e le necessità del nostro Paese.

inusitata, è che un senatore del mio Gruppo è stato allontanato dal seggio elettorale ad operazioni

voluto dagli elettori, l'Italia dei Valori, è fuori dal Consiglio di Presidenza. Questa è una inqualificabile bruttura di cui il Senato si è reso protagonista; è politicamente aberrante e assolutamente vergognoso. Di ciò chiederemo ragione in tutte le sedi politiche.

è entrato nella sala di scrutinio chiedendo di poter assistere allo spoglio dei voti. Dopo aver svolto una consultazione anche con la Presidenza, ci siamo assunti la responsabilità di

Grazie,